Colleghi, tenendo conto delle indicazioni espresse da alcuni Gruppi parlamentari, la Presidenza, apprezzate le circostanze, rinvia la discussione degli argomenti all’ordine del giorno ad altra seduta, che sara` stabilita dalla prossima Conferenza dei Capigruppo.

Io credo, colleghi, che stamani abbiamo fatto un lavoro utile e anche importante, perche´ sono stati approvati provvedimenti rilevanti. Oggi pomeriggio dovevamo affrontare due ratifiche: epero visivamente

Volevo solo rimarcare che nessuno ha affermato che questa mattina non abbiamo fatto un lavoro importante: io ho solo detto che questa mattina abbiamo interrotto anticipatamente l’orario di attivita` di Aula e che avremmo potuto,